in apertura di seduta, ho sollevato alla Presidenza del Senato una questione di indubbia delicatezza, che riguarda un malato gravissimo, Giampiero Steccato di Piacenza, assistito con una miseria da parte dello Stato e della Regione. In apertura di seduta, il Presidente del Senato ha assicurato un intervento dei suoi Uffici affinché il Ministero della salute prenda in considerazione tale questione. Perché intervengo di nuovo, e lo farò fino a che il Ministero non ci darà risposte soddisfacenti? vede, Presidente, nella giornata di ieri, nonostante due interrogazioni da me presentate, nonostante il clamore mediatico e la promessa di intervento da parte della Presidenza del Senato, mi risulta, salvo smentita, che la famiglia di questo malato sia stata convocata dalla ASL e che le sia stato brutalmente detto: non puoi pretendere di più. Ora, stiamo parlando, e vorrei che il Senato ne fosse consapevole, di una malattia che riguarda cinque o sei casi nel nostro Paese, un centinaio in tutto il pianeta.

nuovamente la Presidenza del Senato a pretendere dal Ministero una risposta netta perché non possiamo indurre le persone a desiderare di morire: questo è il rischio che si corre nel caso di Giampiero Steccato.

giustamente e meritoriamente. Posso garantirle che la Presidenza è già intervenuta sia in via informale sia in via formale presso il Governo, anche dopo la sua sollecitazione di ieri, affinché vi sia l'intervento da lei stesso sollecitato. La risposta che ci è stata data è che il Governo si sarebbe mosso entro pochi giorni. Questo è quello che, in questo momento, sono in grado di dirle. La Presidenza del Senato le garantisce che

Presidente, questa estate siamo stati tormentati dagli incendi: la mobilitazione è stata massiccia, ma i danni sono stati ingenti per l'Italia tutta. Da qualche giorno, alcuni quotidiani italiani parlano dell'invenzione di un nostro concittadino, l'ingegnere Pasquale Vurchio, che ha presentato una bomba antincendio per bloccare gli incendi sul nascere.

alla sollecitazione venuta dal senatore Gramazio, ma per un altro aspetto, se lei è così cortese da seguirmi per qualche minuto su una questione che riguarda sempre l'emergenza e, per certi versi, la tragedia degli incendi che ha interessato la nostra penisola per tutta l'estate; estate certamente tra le più calde degli ultimi anni,

anzi, tutt'altro, dal sole potremmo ricavare energia; ma diventa una calamità quando si sviluppano incendi, quando non riusciamo a controllare le situazioni che si determinano sul territorio. Ormai

definire tali coloro i quali appiccano incendi in aree di enorme valore ambientale e naturalistico. quindi parlare di azioni criminali vere e proprie. Il quadro è desolante, Presidente. Le offro pochissimi dati che ho reperito e che risalgono al 30 agosto 2007: 7.164 roghi boschivi; 112.740 ettari, di cui 53.698 soltanto di boschi, sono andati in fumo al 30 agosto. Ferragosto è stato degnamente festeggiato: dal 13 al 19 agosto si sono verificati 636 roghi in tutta Italia. Al primo posto la Calabria

dalle fiamme, nonostante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 luglio 2007 dichiarasse lo stato di emergenza per tutte le Regioni colpite dagli incendi, compresa la Basilicata. Signor Presidente, scusandomi per aver

del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada

subito dopo la fase un po' convulsa della fine dei lavori dell'Aula prima delle ferie, ho notato in merito alle proposte appena varate, di una specie di decalogo il quale, anticipando il decalogo del senatore Calderoli su come evadere le tasse,

che stabilisce l'aggravamento delle ammende, nonché del reato e delle pene, per coloro i quali guidino veicoli in stato di ebbrezza (o comunque con soglia alcolica molto alta) oppure dopo aver assunto sostanze psicotrope. Veniva reso noto che, per come era congegnata la norma, c'era un modo molto singolare di eluderla: dichiararsi talmente ebbri o talmente in preda a cospicue dosi di psicofarmaci o di sostanze psicotrope da non poter nemmeno raggiungere lo strumento con il quale si rileva il tasso alcolico o la presenza nel sangue di sostanze psicotrope.

colpiva il fatto che, in occasione della sentenza relativa ad un gravissimo incidente automobilistico,

di essere in grado di dominare le sbornie mentre si guida l'auto; l'omicidio commesso in queste condizioni è quindi puramente colposo in quanto, quando si è saliti a bordo dell'auto, si aveva la certezza di non incorrere in questa gravissima possibilità. È chiaro che norme che presentano queste caratteristiche non possono essere accettate. Voglio dire però, rispetto alla discussione successiva,

l'effetto di queste notizie è stato quello di introdurre rilevanti ed ulteriori modifiche alle norme del codice della strada in maniera da rendere effettiva la loro incidenza sullo stato di guida e così via. Certo, molto resta ancora da fare. Rapidamente, posso rammentare una norma che ancora c'è e che riguarda i cosiddetti quadricicli.

altra questione molto sentita dalla cittadinanza - che anche con le nuove norme relative agli eccessi di velocità non si mette un argine al fatto che soprattutto alcune amministrazioni locali utilizzano il passaggio attraverso il loro territorio, magari per distanze molto brevi, per intervalli molto brevi, di strade a scorrimento veloce, per impiantare degli *autovelox* allo scopo di fare

derivano da questo tipo di attività debbano essere equamente ripartite tra un fondo sulla sicurezza stradale dell'amministrazione stessa e un fondo sulla sicurezza stradale dello Stato.

che hanno richiesto, tutti, ed ottenuto il carattere di urgenza delle norme da far entrare in vigore

neanche quella dell'esodo estivo, e che i dati sull'incidentalità, letti con un po' più di freddezza, indicano che due terzi degli incidenti, anche per evidenti motivi di congestione dei flussi, e quindi di traffico, si verificano nelle aree urbane

che le misure in materia di sicurezza stradale colgano nel segno di un fenomeno grave che permane sulle nostre strade, fenomeno che presenta dei numeri, una frequenza, una stabilità e degli indicatori assolutamente diffusi sul territorio nazionale,

a fare di più e ad intervenire in particolare sulle aree urbane al fine di attuare il piano della sicurezza stradale approvato nel 1999, ma che è in attesa di risorse e di attuazioni molto più concrete di quelle che siamo stati capaci di realizzare in questi otto

riguardano più aspetti: la guida senza patente, i limiti alla guida di veicoli troppo potenti per i neopatentati, l'inasprimento delle sanzioni e della decurtazione dei punti per il superamento dei limiti di velocità e per l'uso dei telefoni

Signor Presidente, colleghe e colleghi, signor Ministro, il Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea esprimerà voto favorevole sulla conversione in legge del decreto di cui stiamo discutendo, che è il frutto di un confronto di un confronto ampio ed articolato e ha registrato un ampio consenso. In realtà, tutto il complesso di norme che abbiamo discusso è stato il frutto di un ampio e articolato confronto e di un generalizzato consenso, anche grazie (vogliamo ribadirlo come Gruppo di Rifondazione Comunista) alla disponibilità del Ministro che ha lavorato con noi giorno per giorno, fianco a fianco, in Commissione per risolvere i problemi che man mano venivano posti: la discussione è stata sul merito e molto interessante. Il decreto-legge è stata una prima urgente risposta ad una situazione di vera e propria emergenza nazionale: ne abbiamo ampiamente discusso ieri ed è stato ribadito dai colleghi e dallo stesso Ministro in Aula

brevi. Ci convince l'impostazione generale che il Ministro ha sostenuto anche ieri, qui in Aula, poiché riteniamo che un problema così grave, come quello della sicurezza stradale, per essere affrontato in modo adeguato Il risultato complessivo del disegno di legge riteniamo che sia più che accettabile, poiché - secondo noi - sono state arginate

dal disegno di legge che spero riusciremo ad approvare nel più breve tempo possibile. Secondo noi, complessivamente il

relativamente alla sicurezza e al rispetto delle norme, da parte degli autisti, per quanto riguarda il riposo, le pause e così via: ci sembra si tratti di un articolo caratterizzante e importante che recepisce, tra l'altro, le norme europee.

Ritengo importante, ad esempio, essere tornati indietro rispetto al famoso articolo 2, che prevedeva la cosiddetta guida accompagnata a sedici anni, poiché

il ragionamento su una guida consapevole e accompagnata potrà far parte di un decreto legislativo di cui demandiamo al Governo

manifestata e praticata dal Ministro in questa occasione - e che ha significato, per un verso, consentire che il Governo predisponesse un decreto-legge in modo da dare una risposta urgente alle attese dell'opinione pubblica a seguito degli

per misurare, in un confronto aperto, le nostre opinioni. Il decreto è stato utile, a mio modo di vedere; tuttavia, come sapevamo quando si è discusso l'argomento in Commissione, non poteva essere esaustivo, tanto che probabilmente i risultati a livello di riduzione dell'incidentalità

Signor Presidente, il Gruppo dell'Ulivo voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge in esame. È stato molto importante che il Governo abbia assunto questa iniziativa prima

molto distante da quella percepita dalla maggior parte degli automobilisti. In particolare, non si prende atto che in moltissimi luoghi detti limiti non vengono rispettati da nessun automobilista.

presentato riprende un problema molto serio, quello degli accessi stradali nei fondi rustici. Molti si potrebbero domandare cosa c'entrino gli accessi stradali dei fondi rustici: questo problema, collegato a quello della sicurezza, deriva soprattutto da una situazione determinatasi in alcune Regioni (Piemonte e Puglia) a seguito di decisioni dell'ANAS, che hanno portato ad una verifica degli accessi nelle strade di sua competenza, determinando maggiori oneri e canoni per i conduttori dei fondi. Ora, si tratta di intervenire, così come ha chiesto anche il senatore Marcora, per consentire - laddove, in presenza di fondi rustici, vi siano più accessi stradali - il pagamento di un solo accesso stradale, venendo incontro a questa esigenza di sicurezza che non può essere scaricata per i conduttori. Pregherei il ministro Bianchi di tener conto di questa situazione e procedere all'accoglimento di questo emendamento.

quei Comuni che usano i propri impianti semaforici per fare cassa - mi riferisco al famoso *photored* - di dare almeno la possibilità agli automobilisti di individuare visivamente quanti secondi mancano al faticoso rosso!

nuova finestra"). Ho capito la richiesta e la sollecitazione che lei ha rivolto fondamentalmente al Governo. Il ministro Bianchi cortesemente intende risponderle.

di cui dovremo valutare l'entità, prima di mandare avanti un'indicazione del genere; la seconda è che non possiamo immaginare che vi sia una iniziativa non regolamentata in una norma-quadro, di carattere tecnico, per cui si dica quali sono le caratteristiche tecniche dell'impianto semaforico, come avviene per tutti gli impianti di segnalazione, lasciando così il tutto sembrerebbe indeterminato!

hanno lo scopo di adeguare il vigente codice della strada al progresso tecnologico verificatosi nel settore della meccanica agraria, in particolare per quanto riguarda l'aumento delle masse massime delle macchine agricole e della lunghezza massima dei convogli.

contro il parere della Commissione bilancio.

del Ministero delle attività produttive; non è nella totale disponibilità del Ministero dei trasporti prendere un'iniziativa del genere in questa sede. Non siamo pertanto in grado di esprimere parere favorevole.

Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

L'articolo 2 interviene in materia di accertamenti tecnici necessari e di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore. Attualmente è in discussione 10a Commissione il provvedimento di liberalizzazione cosiddetto Bersani-*ter*, sul quale sono stati presentati diversi emendamenti da parte di diversi senatori, che intervengono per assicurare un'apertura del mercato della componentistica auto. Si tratta di un comparto molto importante per il nostro settore produttivo, in cui abbiamo aziende di punta che stanno ottenendo risultati molto importanti anche sui mercati mondiali. Naturalmente, se venissero approvati quegli emendamenti che vanno in quella direzione, in qualche modo si agirebbe anche sulle procedure che qui noi oggi stiamo approvando. Segnalo ciò perché, in caso venissero poi approvati e questo e quello, sarà necessario prevedere una certa correlazione tra i due testi di legge.

chiedo scusa, Presidente,

Il decreto-legge convertito in legge prevede di fatto già l'articolo che viene contenuto nel disegno di legge in approvazione.

contestualmente lo stesso testo di legge. La lettura da dare a questo emendamento è che si applicano le disposizioni dell'articolo 186, al testo di legge già approvato. Nello specifico, il comma 2-*sexies* introduce una fattispecie molto opportuna: infatti, nel caso in cui

alla capacità di guida del conducente e al rispetto delle regole da parte di questo ma anche alla qualità della guida degli altri veicoli, che siano essi autocarri o ciclomotori.

(e spero che l'Aula del Senato voglia essere attenta al tema): «Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena dell'arresto fino a un anno (...)»; «la

che, se si vuole imboccare la strada della sanzione efficace nei confronti di chi guida senza patente, rende la norma completamente sballata. Ricordo che nella fattispecie prevista per l'arresto rispetto alla guida senza patente rientrano non solo il caso del minorenne o del maggiorenne senza patente (soggetti in teoria privi di una preparazione teorica e pratica del mezzo), ma anche tutti coloro ai quali la patente è stata ritirata.

Chiedo di poter sopprimere l'ultimo periodo, perché mentre posso comprendere l'esigenza che viene rappresentata nella stesura dell'articolo, del comma che viene proposto, ritengo francamente che esso rischi di andare in stridente contraddizione con quanto si è sostenuto nell'affermare

così dire, non minima (un anno di arresto), per cui indubbiamente vi è un comportamento consapevole da parte del reo, ma credo che si possa consentire la possibilità, appunto, di una recidiva nell'arco di un biennio. Esprimo pertanto parere contrario

di una sanzione o di una pena corrispondente ad un reato si tratta di trovare l'equilibrio tra la gravità e la sanzione. In questo caso

domani mi presento senza patente, dopodomani, se lo faccio di nuovo, scatta l'arresto fino ad un anno e questa recidiva è valida nell'arco di due anni. Mi sembra una sanzione sufficientemente equilibrata rispetto all'infrazione.

È da qualche settimana che apriamo giornali e vediamo quale fuoco di fila viene addosso alla politica, dica che l'antipolitica sta prendendo il posto nostro. Non è solo un fatto di costume, è anche un fatto di contenuti: più leggi sciocche, incomprensibili

Non è possibile - e vado a sostenere l'emendamento del senatore Storace - che si punisca in modo più grave chi la patente ce l'ha

Un abilitato, cioè, viene condannato ad una pena pecuniaria e all'arresto e non chi guida senza patente in quanto inabilitato. Quando l'abbiamo detto noi sembrava che si volesse punire tutti i disgraziati provenienti dall'estero, senza che salgano su una macchina e combinino tutto quello che combinano. Il problema è dell'abilitazione: non c'è congruenza nella sanzione tra chi viola una norma di comportamento alla guida rispetto a chi non ha mai ottenuto una patente. Un'altro punto altrettanto incongruente non è possibile paragonare alla stessa stregua chi la patente non l'ha mai ottenuta da chi distrattamente se l'è lasciata scadere in tasca, ma che avrebbe potuto

Più leggi sciocche faremo in questo senso, più avremo l'opinione pubblica che dirà: andate a casa, fatevi sostituire. Insomma, signori, Ministro, un minimo di attenzione nel seguire una scala di valori

e la trasformazione in un subemendamento all'emendamento del relatore. Lo dico perché l'argomento che stiamo discutendo è piuttosto rilevante e delicato; lo dico per consapevolezza delle decisioni che stiamo assumendo. Ha facoltà

Ora vorrei che vi fosse un po' di libertà nella discussione. Vorrei che il Senato, anche in ragione delle considerazioni svolte dal senatore Di Lello (notoriamente è difficile che io ci possa andare d'accordo, ma c'è qualche momento in cui ci si ispira al buonsenso),

entro il quale sarebbe entrata in vigore. Posso capire le ragioni del Ministro che dice: prima era depenalizzato, poi lo introduciamo come reato, adesso arriviamo all'arresto; non possiamo esagerare. Questo mi sembra il senso del ragionamento del Ministro, apprezzabile da un certo punto di vista. Però vi chiedo se una sanzione che viene prevista e poi non è efficace non ci esponga a critiche enormi da parte di tutti. Sarebbe una questione che non capirebbe nessuno.

per chi intende guidare i motocicli. Voglio semplicemente sottolineare che l'emendamento 4.800 si propone di assimilare i quadricicli ai motocicli per quanto riguarda le prescrizioni per la loro guida. Ricordo che per "quadricicli leggeri" si intendono comunemente le cosiddette vetturette, quelle che hanno una massa a vuoto inferiori a 350

Signor Presidente, cercherò di essere sintetico perché le motivazioni sono molte. L'articolo in esame, combinato con l'articolo che tratta lo stesso argomento del decreto‑legge che purtroppo, inopinatamente

conseguimento della patente non si possono guidare veicoli al di sopra di una certa potenza. Il primo e principale vizio di questo articolo, come ha già molto ben detto nella discussione generale il senatore Cicolani,

in questo modo obblighiamo le famiglie all'acquisto di un'auto apposta per il neopatentato; diversamente, il neopatentato nella maggior parte dei casi dovrà rimandare il tempo in cui potrà guidare, sia pure solo ogni tanto,

possibile guidare. Il Ministro in un colloquio privato ha detto che la "500" è inclusa: ho motivo di credere che lo dica fondatamente, ma i dati che io trovo sui giornali specializzati dicono che, facendo il semplice rapporto tra potenza in kilowatt kilowatt e la massa di questi veicoli, si ha una potenza da poco ad un po' più di poco superiore ai 55 kilowatt per tonnellata, per cui la maggior parte dei modelli non può essere guidata. Allora, se un diciottenne ha la fortuna di avere dei genitori che hanno la possibilità di acquistare

a 21. Il Partito Democratico dà la possibilità di votare alle elezioni primarie a 16 anni, il sedicenne può decidere chi si candida, quanto meno, a guidare il Paese, ma non può guidare un'automobile: mi sembra esagerato. Allora, capisco la prudenza, ma come ho già detto ieri si tratta di norme elaborate con il massimo delle buone intenzioni però nei fatti discriminano le famiglie che hanno determinate possibilità da quelle che non le hanno. La norma che fa entrare in vigore questo limite a partire dalle patenti conseguite sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge ha poi la seguente conseguenza: coloro che hanno già conseguito la parente oggi, con un esame e con un addestramento che non è aggiornato, dunque non è reso più severo ed accurato dalle norme che il disegno di legge in esame introduce, cioè chi ha una patente che dovrebbe essere meno valida, può guidare qualunque automobile; la conseguirà fra sette mesi, cioè con corsi ed esami più accurati, potrà guidare solo le macchinette, possibilmente se qualcuno gliele compra.

e, con l'emendamento 5.802, di andare più sulla prevenzione e sull'educazione prevedendo

l'emendamento 5.803 prevede che i giovani possano guidare una macchina di più alta cilindrata se accompagnati dai genitori oppure da un adulto che abbia la patente almeno da dieci anni, in modo da essere assistiti nella guida. Presidente, colleghi, anche se l'Aula è un po' distratta, vorrei che assumesse consapevolezza di che cosa stiamo per approvare, perché all'interno di questo provvedimento, complessivamente ragionevole e positivo, resta uno degli elementi assolutamente negativi e che verrà in tal modo percepito

è andato ad abitare in periferia o in campagna), deve prendere la patente, anche se ha 40 anni o 35, per i primi tre anni

requisiti previsti li rispettava soltanto ed esclusivamente la "Panda", tanto per capire di cosa parliamo. Nella attuale formulazione sembri che rientri anche la nuova "500".

luogo, veramente mettiamo in discussione le pari opportunità in questo caso del nostro Paese? Veramente tutte le famiglie hanno la possibilità di acquistare una macchina per un neopatentato? La macchina media delle famiglie che hanno un solo veicolo è una nuova "500", una o piuttosto non è una macchina che ha una potenza leggermente superiore, in grado di essere utilizzata per varie funzioni? Si rientra certamente nel secondo caso. Noi non diamo quindi la possibilità alle famiglie meno abbienti

a coltivare i terreni. Immaginate quelli che il sabato o la domenica vanno con la *jeep* in campagna o quelli che ci vanno tutti i giorni. Le *jeep* non rientrano in questa previsione normativa, ma si tratta di mezzi che servono per lavorare. Pensate che discriminazione andiamo ad introdurre nel nostro Paese!

non è giusta l'equazione «minore potenza, maggiore sicurezza» (semmai «minore velocità, maggiore sicurezza»). Ancora di più, in questa maniera, obbligando chi può permetterselo ad avere un altro veicolo, si aumenta il parco circolante nel nostro Paese, che è certamente causa non ultima fra quelle che

di sopprimere l'articolo in esame e, semmai, di prevederlo nella delega, visto che quella prevista all'articolo 29 contiene tutte le norme relative alle patenti di guida. Pensate anche a come sia facile eludere quest'articolo, perché basta che un neopatentato prenda la patente C

inutile, che va nella direzione opposta a quella della sicurezza stradale e si rivolge in maniera estremamente negativa alle famiglie più deboli del nostro Paese.

preme prima sviluppare una riflessione di carattere generale, perché mi sembra che il tema trattato dall'articolo 5 sia particolarmente avvertito e sentito, come hanno illustrato i presentatori degli emendamenti. verrebbe da dire, riprendendo lo *slogan* d'effetto di una pubblicità di successo, che la potenza senza controllo è nulla, per affermare sostanzialmente che è sul controllo che dovremmo probabilmente appuntare ed addensare la maggiore attenzione.

Pertanto, l'elemento di limitazione della potenza, che in molti casi consente velocità davvero eccessive, è stato ritenuto comunque un elemento di taratura abbastanza adeguato. Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, riteniamo che la riformulazione operata dal Governo con l'emendamento 5.500 in qualche modo consenta davvero un equilibrio, che garantisce - ovviamente rispetto a prestazioni eccessive da parte degli autoveicoli

l'altro parametro dei 70 kilowatt assoluti, che ovviamente tende a tarare la potenza in funzione della velocità, chiaramente per le macchine di maggiore stazza. Pertanto, sostanzialmente, accoglieremo

riflessione è che i centri di guida sicura, purtroppo, non sono una realtà estesa in tutto il Paese: questo, quindi, non può essere un elemento di riferimento valido; del resto, anche tra quelli presenti,

Signor Presidente, vorrei spiegare brevemente qual è la *ratio* che ha condotto a presentare l'articolo che prevede limitazioni nella guida di alcuni autoveicoli per i neopatentati. Faccio presente che questa norma è stata d'iniziativa governativa fin dall'inizio, fin dalla presentazione del disegno di legge alla Camera.

ci ha portati alla considerazione, che a me sembra molto sensata, per cui una persona, quale che essa sia - è stato detto potrebbe non essere un giovane, ma sta di fatto che la stragrande parte di quelli che conseguono la patente la prima volta è un giovane di 18 anni - non è, per il grado di abilità che ha conseguito,

Detto questo, abbiamo provato a capire quale fosse la soglia dei veicoli da rendere disponibili e si era fissata in un primo tempo in 60 kilowatt per tonnellata. Faccio presente quindi che non è solo la potenza del veicolo, ma la potenza rapportata al peso: evidentemente un veicolo molto pesante

anche per l'evoluzione tecnologica che vi è stata in questi ultimi anni, grandi prestazioni, in termini sia di velocità, sia di accelerazione e quant'altro. Quindi abbiamo proposto una riduzione che forse - qui, debbo ammettere un po' frettolosamente - nel decreto di fine luglio è diventata di kilowatt per tonnellata, rispetto alla quale ci è stato fatto notare che veniva esclusa una gamma molto ampia, forse eccessiva, di veicoli, ivi comprese quelle auto che sono state citate, come la 500 o altro, la Toyota Yaris, e via dicendo. A questo punto, abbiamo affidato agli uffici tecnici del Ministero uno studio che, appunto, partito alla fine di luglio e completato poche settimane fa, tendesse a trovare un equilibrio accettabile per questa limitazione. La proposta che qui abbiamo avanzato, ossia del tetto di 55 kilowatt per tonnellata,

Cito i casi della Peugeot 207, della Citroën C4 e della 500. Restano escluse - questo vorrei sottolineare - dalla possibilità di guida tutte le monovolume medio-grandi, tutti i SUV, i veicoli a velocità elevata tipo Tuareg, Passat, Alfa 159 e così via.

che in direzione di assicurare maggiori livelli di sicurezza sulla strada, limitare l'uso di veicoli molto potenti ai giovani neopatentati sia uno degli aspetti basilari.

Vorrei ricordare un dato. Il Ministro, con la sua grande cortesia, di cui lo ringrazio, ci ha detto che la determinazione di 55 kilowatt per tonnellata è frutto di uno studio di settimane degli uffici del Ministero.

poi c'è la tassa di circolazione e poi, se si vuole anche guidare l'auto, bisognerà metterci la benzina e fare la manutenzione, possibilmente spesso. Si è parlato tanto delle famiglie che non arrivano alla fine del mese, e pensiamo che spendere 3.000 euro solo per iniziare a guidare un'auto sia una spesa da poco. Ripeto, il subemendamento in esame almeno rimedia parzialmente a questo problema. Non dobbiamo discriminare fra le famiglie, che possono comprare un'auto apposta per un diciottenne e quelle che non possono, e non dobbiamo neanche fare una discriminazione all'incontrario per cui chi consegue la patente oggi, con le norme attualmente in vigore, potrà guidare guidare qualunque auto e, chi invece consegue la patente tra sei mesi, quando ci saranno esami più severi ed esercitazioni più accurate, potrà guidare solo le macchinette. Francamente, ciò va veramente contro ogni logica.

Signor Presidente, vorrei per un attimo ritornare sul tema della 500. Ho detto che se ne sono occupati gli uffici; ovviamente mi assumo tutte le responsabilità, nel caso avessero sbagliato. Leggendo testualmente dalla relazione che mi è stata consegnata, risulta che dalla verifica è risultato che il nuovo valore

al parco veicoli conducibili dai neopatentati vetture quali, ad esempio, la Fiat 500, la Toyota Yaris e simili.

Presidente, con l'emendamento 7.2 poniamo un problema. Dovendo richiedere alle autoscuole nuove e vecchie maggiore professionalità, e per far diventare queste aziende dei veri e propri centri di formazione per i conducenti, si rende necessario prevedere che tutte le autoscuole debbano essere attrezzate e formate per offrire alla clientela ogni tipo di servizio. Oggi, infatti, si sta verificando che molte autoscuole aprono chiedendo di essere ricomprese nel tipo B «Insegnamento limitato alle sole patenti A e B» e quelle esistenti, per adeguarsi alla logica della concorrenza, chiedono di poter svolgere solo insegnamento limitato. Tutto ciò fa diminuire la quantità di servizi offerti, a discapito dell'utenza che ha difficoltà a trovare autoscuole che possano formare al conseguimento di patenti superiori. Inoltre, le poche scuole o consorzi attrezzati per

14, la richiesta è dettata dal fatto che dovendo prevedere intensi e seri percorsi formativi per chi accede alla professione di istruttore e di insegnante, non è concepibile prevedere che come le autoscuole esistenti possa svolgere questi corsi. Occorre prevedere che solo le associazioni delle autoscuole, che sono già attrezzate per lo svolgimento di corsi altamente professionali, possano organizzare questi corsi obbligatori con la collaborazione magari di università e di docenti esterni. Per tali ragioni sollecito il rappresentante del Governo e il relatore a tenere conto

del Governo è conforme a quello del relatore. Aggiungo che si tratta di modifiche regolamentari, che quindi non necessitano di una norma primaria e che, in ragione della legge Bersani, il Ministero dei trasporti sta già predisponendo un decreto

sull'emendamento 8.2 il parere è contrario in quanto è inopportuno dilatare ulteriormente i tempi per il proprietario del veicolo, dal momento che la dilatazione dei tempi consente l'intensificazione di un fenomeno già presente,

Per questo c'è anche la necessità di comprendere se questi rilevatori siano attivi o no: il più delle volte non sono attivi e ciò comporta che l'automobilista tenta, passa, o non passa, e poi magari si ritrova multato.

che, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individuano le stesse tratte e autorizzano la collocazione. Pertanto, una previsione

Mi permetto poi di insistere anche perché la mia proposta va nel senso della tutela della salute, soprattutto dei minori. Molte volte abbiamo visto maggiorenni fumare in presenza di bambini, anche neonati. Cerchiamo allora di avere un po' di considerazione e di coraggio per limitare questo danno che viene procurato ai nostri figli. Chiedo,

a modificare le percentuali in misurazioni di tempo effettivo, in minuti, per poter rendere più chiara la norma.

Il tema trattato all'articolo 14, riguardante la disciplina di guida dei veicoli adibiti al trasporto di persone e cose, è stato particolarmente dibattuto in Commissione. Tra l'altro, l'articolato è il frutto di un accordo con la categoria a seguito di una trattativa molto complessa e delicata. Noi riteniamo che l'emendamento proposto dal Governo abbia accolto, per quanto parzialmente, in maniera sufficientemente adeguata le motivazioni di buon senso che sono state - devo dirlo - sinceramente esposte dal presentatore dell'emendamento

ampiamente discusso in Commissione. Ricordo il tema: si tratta di stabilire che la guida dei mezzi pesanti, generalmente conosciuti come TIR, viene regolamentata da opportuni periodi di sosta e di riposo.

Il Senato è in numero legale, nonostante le apparenze.